Occorre procedere all’avvicendamento fra un componente effettivo e un componente supplente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa-UEO. Come giacomunicato per le vie brevi ai Gruppi, la Presidenza si avvarra a tal fine della procedura prevista dall’articolo 25, comma 5, del Regolamento, costantemente applicata. Se non si fanno osservazioni, cosırimane stabilito. Sulla base delle designazioni del Gruppo interessato, il senatore Sinisi e la senatrice Soliani – entrambi gia facenti parte della delegazione – sono pertanto nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente. Onorevoli colleghi, comunico che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto ieri alla Camera dei deputati la questione di fiducia sull’approvazione, senza ulteriori modifiche rispetto al testo giaapprovato dal Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale. Il Senato tornera pertanto a riunirsi, come giastabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, martedı 19 settembre, alle ore 17, per il seguito dell’esame del disegno di legge n. 635,